L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'università e della ricerca.

Signor Presidente, signor Ministro, che la riforma del servizio taxi voluta da questo Governo non stia funzionando è evidente ogni volta che si scende nella bellissima stazione stazione della città di Roma o in qualsiasi altra città; pensiamo a Milano dove in questo periodo c'è il Salone del mobile: code code allucinanti che non sono degne di un Paese civile. Lei ci dirà che sono i sindaci che devono operare. Sì, è molto facile fare scaricabarile. Di fatto, la riforma non ha funzionato per le stesse parole dette dalla ministra Santanchè, sconsolata, di fronte ad una coda taxi alla stazione Termini. Invece di incrementare non solo le licenze, e quindi magari risolvere il problema dei taxi, ma anche la possibilità di scelta, stranamente questo Governo ha deciso di infierire sul noleggio con conducente, aggravando la normativa, mettendo ulteriori balzelli burocratici, e soprattutto facendo rispettare l'obbligo di fermata con ritorno in autorimessa, cosa che non è mai avvenuta, nonostante la Corte di giustizia europea abbia detto più di una volta che la normativa italiana è assolutamente anticoncorrenziale, perché è evidente

obbligatorio - oltre che degno di un Paese civile - togliere tutti i balzelli burocratici e consentire una libera concorrenza,

ringrazio la senatrice interrogante perché il Governo intende fare quello che i passati Governi non hanno fatto per anni e non certo, ovviamente, penalizzare lavoratrici, lavoratori e imprese dei noleggi con conducente a esclusivo vantaggio dei taxi, come si afferma nelle premesse. Questo non è interesse né mio, né di nessun altro, visto che stiamo lavorando per l'interesse dei consumatori e - come ha detto lei - i sindaci adesso hanno la facoltà di mettere sul mercato nuove licenze taxi e, da autonomista, sono convinto che faranno il meglio. Taxi e NCC sono due servizi diversi e complementari e solo valorizzandoli entrambi potremo offrire ai cittadini un trasporto alternativo a quello di linea - su cui peraltro stiamo investendo miliardi di euro - efficiente e di qualità. Abbiamo già fatto - ne ho presiedute personalmente diverse - delle riunioni insieme al Ministro delle imprese e al Ministro dell'interno; stiamo lavorando con le categorie per sbloccare tre decreti attuativi che le categorie attendono da anni. Abbiamo avuto sei incontri; le bozze dei tre decreti sono state illustrate e discusse e abbiamo ricevuto più di 400 osservazioni dalle categorie. Il lavoro è faticoso e doveroso per diversi motivi. Il primo è che il registro informatico nazionale di taxi e NCC consentirà di sbloccare il rilascio di nuove autorizzazioni NCC, superando uno stallo che dura da sei anni, anni, come lei auspicava. Il secondo è che grazie a questi decreti potremo conoscere il numero reale degli operanti nel settore che ad oggi è sconosciuto. Il terzo è che la digitalizzazione delle procedure a superare la trasmissione cartacea che nel 2024 ovviamente non è compatibile con le esigenze dell'operatore e dell'utente. Il quarto dare attuazione alla legislazione vigente che regola taxi e NCC al fine di garantire che i servizi rispondano a precisi obiettivi pubblici, compresa la capillarità sul territorio, non solo nelle grandi città. e più importante fra gli altri motivi è l'esigenza di garantire la regolarità nello svolgimento dei servizi di trasporto non di linea contro ogni forma di abusivismo. Su questi punti confermo l'intenzione di risolvere il problema delle sanzioni per gli NCC come atteso dalla categoria, che andranno allineate a quelle dei taxi e differenziate in base alla gravità della condotta. L'obiettivo è di veicolare questa modifica (articolo 85) d'intesa con il ministro Urso già nel prossimo disegno di legge sulla concorrenza. Confermo che i decreti non prevedono alcun lasso di tempo obbligato o alcuna pausa tra una corsa e l'altra per gli NCC; anzi, abbiamo cercato di favorire la continuità nello svolgimento del servizio, evitando il ritorno in rimessa in tutti i casi in cui vi siano più servizi collegati. In conclusione, è evidente che la digitalizzazione consentirà di combattere il *far west* dei comportamenti che si sono stratificati nel tempo a causa dell'inattuazione della legge quadro di settore. L'obiettivo comune è superare la conflittualità

vorrei rinfrescare la memoria al ministro Salvini: durante il Governo Conte I lei aveva un vice Ministro che si chiama Edoardo Rixi;

avete governato più di qualsiasi altra forza politica che siede in questo Parlamento il Ministero dei trasporti, a cui ovviamente bisogna collegare il suo arrivo da Ministro e di nuovo quello del vice ministro Rixi.

I risultati sono che voi avete elaborato una strategia per la quale, sostanzialmente, le licenze nuove ai taxi non le date perché dovete salvaguardare la categoria dei taxi. Basta farsi un giro, Ministro, perché la realtà prende sempre il sopravvento sull'immaginazione, anche la sua. Basta farsi un giro in città: le persone rimangono a piedi, non hanno il servizio semplicemente perché i taxi non ci sono. Basta fare una cosa: aumentare quelle licenze, dare la possibilità che aumentino. Lei questo non lo vuole perché quella è una categoria alla quale lei tiene particolarmente, immagina di differenziare sanzioni, penalizzando il noleggio con conducente; immagina un'identificazione di chi viene trasportato, che è differente e va anche a ledere il principio della *privacy*; immagina il ritorno in rimessa, cioè delle norme a dir poco assurde nei confronti di una categoria che dovrebbe - quella sì - chiamare il tribunale dei diritti umani. umani. Sostanzialmente, lei sta mettendo in atto delle attività di carattere persecutorio nei confronti del noleggio con conducente. Il problema vero non è per quale motivo lei ce l'ha particolarmente con la categoria degli NCC e vede così favorevolmente la categoria dei taxi. Il problema vero è che lei sta immobilizzando

- come le ho confermato e dimostrato - in questi anni ha governato attraverso i suoi uomini tantissimo questo Ministero, secondo me una domanda su quanto efficace siano state le sue politiche probabilmente se la dovrebbe porre. Di certo oggi non ha più alibi: lì ci siede lei, è lei il Ministro dei trasporti; Edoardo Rixi è il vice ministro dei trasporti, sempre della Lega; Roma è completamente nel caos, Milano molto spesso è nel caos. Si metta una mano alla coscienza: non dico di preferire o far prevalere l'interesse sugli NCC, ma almeno cerchi di aumentare qualche licenza per i taxi e di dare un minimo di giustizia a questa politica che - ripeto - nei confronti di una categoria ha dei tratti di vera e propria persecuzione.

premetto che nel marzo del 2023 abbiamo preso atto del decreto-legge che sancisce la sua volontà di realizzare il Ponte sullo Stretto e attraverso il decreto è evidente che vuole farlo in fretta. Abbiamo visto che nella legge di bilancio ha stanziato 11 miliardi dei 14 probabilmente necessari, a nostro avviso ipotecando così un Ministero e addirittura chiedendo aiuto alle Regioni dal Fondo di sviluppo e coesione, le Regioni Sicilia e Calabria. bisogna considerare che il progetto sembra ricalcare quello del 2011, quindi è un progetto vecchio; che nel progetto presentato non c'è un elaborato di stima economica, e quindi in realtà non sappiamo ancora quanto costerà la realizzazione del Ponte considerare le 239 richieste di integrazione della commissione VIA-VAS. Signor Ministro - per usare un termine suo - sono non bruscolini, ma integrazioni importanti: per esempio, studio di impatto ambientale; studi sugli scenari sismici e di maremoto; elaborati di morfodinamica costiera; non ultimo, l'impatto di acque superficiali e sotterranee, perché il progetto, così come è scritto, rischia di lasciare Messina senz'acqua durante la realizzazione del Ponte. Inoltre, anche il Ministero della cultura (quindi non il MoVimento 5 Stelle) chiede ulteriori integrazioni, perché prende atto che il progetto è vecchio e chiede integrazioni significative alla documentazione paesaggistica e archeologica (leggendo dal documento si evincono le parole «carente», «insoddisfacente», «non sufficientemente approfondita»). Noi le chiediamo, signor Ministro, intanto se lei è a conoscenza, volendo realizzare il Ponte, un'opera mastodontica, che il progetto è vecchio, carente, approssimativo e sommario e, per questo, pericoloso. Le chiediamo se è a conoscenza che, per realizzare bene un'opera, che lei dice verranno da tutto il mondo a vedere, è necessario dare il tempo dovuto a chi deve realizzare gli approfondimenti. Le chiediamo: non è forse opportuno rivedere o riconsiderare l'opera per il bene dei cittadini, anche perché andiamo a spendere risorse importanti dei cittadini? A noi, infatti, viene un dubbio. Tutta questa corsa è perché lei vuole realizzare un Ponte che però, con questo progetto, non starebbe in piedi? O sta correndo verso le elezioni europee?

il Ponte lo faranno i migliori tecnici italiani, giapponesi, danesi, spagnoli e americani. In base a quello che l'interrogante chiedeva, il documento prodotto dalla commissione VIA lo scorso 15 aprile rientra nelle attività ordinarie previste per qualsiasi progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale. Non rappresenta assolutamente una bocciatura del progetto. Anzi, il Ministero dell'ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA, avanzando, giustamente, richiesta di integrazioni documentali istruttorie in linea con le procedure per opere assimilabili. La bontà del progetto non viene messa in discussione: progetto, peraltro, approvato all'unanimità dal Comitato tecnico scientifico composto da alcuni dei docenti universitari delle migliori università in discussione l'elevatissimo livello scientifico ingegneristico degli studi condotti. Stiamo parlando di un progetto strategico che, insieme ai 30 miliardi per il miglioramento delle strade, autostrade e ferrovie in Sicilia e agli altrettanti in Calabria, darà lavoro, sviluppo e speranza a due delle terre col più alto tasso, ahimè, di disoccupazione giovanile dell'intera Europa. Il progetto prevede un ponte sospeso a campata unica di 3.300 metri. Per un progetto di tale complessità, per il quale la società proponente, che ha confermato l'obiettivo di aprire i cantieri entro l'estate, ha inviato circa 10.000 elaborati, non può stupire che la commissione richieda approfondimenti di dettaglio. La richiesta di integrazioni nell'ambito della valutazione di impatto ambientale per progetti infrastrutturali è del tutto fisiologica. Per progetti di complessità tecnica e valore di investimento di molto inferiori rispetto al progetto del Ponte le richieste di integrazioni formulate dalla commissione VIA arrivano anche al centinaio. Per quanto detto, il numero ed il contenuto delle osservazioni non desta preoccupazione ai tecnici che ho interpellato. La società Stretto di Messina ha comunicato che le integrazioni richieste saranno fornite entro i termini previsti, ovverosia giorni. Aggiungo, inoltre, che lo scorso 16 aprile, quindi questa settimana, si è tenuta la prima riunione della Conferenza di servizi istruttoria. Alla riunione di insediamento hanno partecipato la società Stretto di Messina e rappresentanti dei Comuni dell'area, dell'Autorità portuale e delle amministrazioni coinvolte. Dopo la presentazione del progetto, è stata così avviata la fase istruttoria, che arriverà all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPESS. Questi dati sono la dimostrazione che l'intero procedimento prosegue con l'opportuna celerità e con ogni attenzione possibile, nella consapevolezza che, insieme a tutte le altre opere che attendevano da anni di essere cantierate su strade, autostrade e ferrovie, in Sicilia e in Calabria, il Ponte sullo Stretto sarà un'opera utile,

che le critiche e le osservazioni (più osservazioni che critiche) fatte nel contesto di analisi della valutazione d'impatto ambientale, sono ambientale, sono osservazioni che non si vedono normalmente a progetti anche di caratura decisamente inferiore rispetto a questa, che è una imponentissima opera pubblica, di un valore economico rilevantissimo e anche di grande complessità tecnica. Gli ingegneri non faranno il Ponte. Gli ingegneri lo progettano: a realizzarlo sarà qualcun altro. La parte progettuale che oggi abbiamo davanti è una progettazione lacunosa, dove vengono richieste integrazioni su aspetti sismici che dovrebbero essere parte integrante ed immediata di un progetto serio. D'altra parte, lei, nel 2016, diceva che non era convinto di fare un Ponte che, le dicevano, potrebbe crollare. Quindi, evidentemente anche da parte sua vi era qualche preoccupazione.

parta quest'estate. Potranno partire, forse, l'accantieramento e le opere propedeutiche all'accantieramento. Ma questo non significa che partano i lavori per il progetto del Ponte. E viste le osservazioni della Commissione, credo che non sarà neanche questa estate. Però, al netto della posizione nel merito dell'opera, io credo, in modo molto pragmatico, che sulle opere pubbliche non ci possa essere un "no" aprioristico e nemmeno un "sì" aprioristico; le opere pubbliche che servono vanno realizzate e bisogna trovare la scala di priorità.

e il contrario di tutto quotidianamente), se vuole realizzare quel Ponte, signor Ministro, la prego, non ne parli più, perché fa perdere di credibilità anche a una mera opera pubblica.

Signor Ministro, quelli della casa, dell'edilizia e dell'emergenza abitativa sono argomenti che hanno assunto nel tempo un'importanza significativa per il Paese. Moltissimi sono i cittadini che tentano da anni di porre rimedio a situazioni di leggera irregolarità del proprio immobile, spesso viziato da difformità edilizie lievi e non sostanziali, attendendo da troppo tempo risposte certe. Spesso si tratta di difformità sul proprio immobile di cui gli stessi proprietari sono incolpevoli, se non addirittura ignari, soprattutto per gli immobili edificati da altri

non consente di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi casi; tale situazione comporta inoltre un consistente aggravio amministrativo a carico degli uffici delle amministrazioni comunali competenti che, a causa della frammentarietà della della disciplina di settore, non riescono a fornire risposte in tempi certi alle richieste di accertamento dello stato legittimo dell'immobile, limitandone la commerciabilità, con ripercussioni severe l'esecuzione di interventi di semplice manutenzione ordinaria, di messa in sicurezza o di efficientamento energetico degli edifici. Le chiedo quali iniziative intende adottare al fine di adeguare la normativa in materia edilizia alle attuali esigenze degli operatori del settore e di risolvere quindi il problema

ringrazio la senatrice Minasi della Lega, che mi permette di dare risposta a questa Assemblea, ovviamente, e a chi è a casa nello stesso tempo, perché il tema casa e le difformità interne alle quattro mura domestiche riguardano - secondo una stima dell'Ordine degli ingegneri - ben più della metà delle case

la veranda, la finestra spostata di 20 centimetri rispetto alla piantina originaria di quant'anni prima. Noi viviamo tutti in condomini o in abitazioni singole: case che hanno subito ristrutturazioni negli anni, a carico dei precedenti proprietari, del nonno, del genitore, dell'eredità. L'obiettivo di oggi, come abbiamo illustrato a tutti gli operatori, dopo numerose riunioni sul piano casa, è di arrivare entro la fine di maggio all'esame di quest'Aula del Parlamento con alcune modifiche che riguardano - ripeto - non gli abusi esterni, ma tutto quello che c'è all'interno delle quattro mura: difformità formali legate alle incertezze interpretative, che per tanti immobili bloccano la possibilità di vendere o comprare casa; difformità edilizie interne alle case, ovvero quelle modifiche derivanti da manutenzione ordinaria o straordinaria, che attengono alla disciplina delle tolleranze costruttive, di cui aumenteremo la percentuale; difformità che potevano essere sanate all'epoca di realizzazione, ma non più sanabili oggi, a causa della disciplina della doppia conformità. Stiamo inoltre intervenendo sulla possibilità di ampliare i cambi di destinazione d'uso per rendere più agevoli le variazioni di utilizzo di una unità immobiliare o di un immobile. Tutto questo per liberare gli uffici comunali da milioni di pratiche, per incassare quello che i cittadini vogliono poter pagare, pur di tornare totalmente padroni del loro bene. Si tratta nel complesso, quindi, non di un condono per chi ha costruito la villa in riva al mare, lungo il fiume, in aree protette architettonicamente o idrogeologicamente pericolose se uno ha la cameretta per il secondo figlio ereditata dal nonno o dal genitore, penso sia più utile che paghi al Comune una quantità di denaro per poter tornare tranquillamente in possesso della propria abitazione - con l'obiettivo finale di diminuire il costo degli affitti. se si riportano sul mercato milioni di immobili che oggi sono bloccati, si fa un buon servizio alla pubblica amministrazione e si arriva ad abbassare il costo degli affitti, soprattutto nelle grandi città. L'impegno entro maggio è che questo lavoro che stiamo portando avanti da un anno e mezzo - unico Governo che se n'è fatto carico - diventi realtà.

relativo al patrimonio immobiliare sia importantissimo per il nostro Paese, perché l'Italia ha un immenso patrimonio immobiliare di proprietà dei cittadini, il cui valore nel 2022 ammontava a 5 miliardi di euro, che sono quasi tre volte il nostro PIL. Oggi il 70 per cento delle famiglie vive in una casa di proprietà e si trova spesso ad affrontare questi problemi che le normative attuali e la burocrazia non aiutano a risolvere. piccoli problemi - come lei, signor Ministro, ha detto - che non costituiscono abusi edilizi, ma hanno pesanti conseguenze se non permettiamo di regolarizzare sulla commerciabilità dell'immobile, sulla loro fruibilità e anche sugli uffici amministrativi. Signor Ministro, crediamo che la sua politica di sburocratizzazione e velocizzazione delle procedure sia senz'altro la soluzione da seguire. Ciò significa dare fiato all'edilizia, al settore immobiliare e aiutare le famiglie anche ad alleggerirsi da pensieri ed ansie legate a queste irregolarità. Significa altresì rendere più fruibile il mercato immobiliare, sempre nel rispetto massimo della sicurezza e della legalità, che sono contrastate dall'opposizione unicamente sulla base di pregiudizi ideologici che certamente non sono nell'interesse della collettività. La ringrazio ancora per il suo impegno e per il lavoro condotto peraltro sulla base dell'ascolto degli operatori di settore e quindi certamente centrato sulle migliori soluzioni possibili.

dall'11 al 13 aprile si è tenuto a Milano, nella sede di Palazzo Reale, la riunione dei Ministri del G7 trasporti presieduta dall'Italia, cui hanno partecipato, oltre all'Unione europea rappresentata dalla Commissaria ai trasporti, le delegazioni dei Ministeri di infrastrutture e trasporti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Il vertice che si è tenuto nel capoluogo lombardo è stato anche l'occasione per chiarire e comprendere le modalità con cui le Nazioni del G7, alla luce della crescente instabilità globale, intendono affrontare le sfide del futuro della mobilità. Segnatamente, l'attenzione è stata posta sull'esigenza di rafforzare i sistemi di trasporto in caso di eventi estremi e imprevisti, come ad esempio le le crescenti tensioni geopolitiche, il cambiamento climatico o gli attacchi informatici, creando e rafforzando strumenti di coordinamento e cooperazione a livello del G7. Tra i temi affrontati, l'adeguamento del settore dell'*automotive* alle criticità ambientali è stato oggetto di un profondo e prolungato confronto tra i partecipanti, culminato nell'unanime consapevolezza di non poter considerare come unica soluzione al problema la trasformazione in elettrico degli attuali veicoli a motore, pubblici e privati, ritenendo, per contro, necessario concentrarsi sullo sviluppo di biocarburanti capaci di salvare le filiere del motore endotermico. Con la presente interrogazione si chiede di sapere quali iniziative in seguito a quanto emerso dal G7 dei Ministri dei trasporti, per conseguire il passaggio da una transizione ambientale semplicemente ideologica ad una pragmatica ed economicamente sostenibile.

ecologica e non ideologica, che non passi dal "tutto subito, solo elettrico", che sarebbe solo un enorme regalo alla Cina. Rischiamo di passare dalla dipendenza dal gas russo a quella dall'elettrico cinese: dobbiamo superare questa follia, che non ha alcun senso ambientale ed economico. La dichiarazione finale, approvata da tutti i Ministri del G7, peraltro parla proprio di neutralità tecnologica, quindi superando l'ideologia imposta dai Timmermans e dalla sinistra al Parlamento europeo e in Commissione europea. È un testo che getta le basi per un G7 che guarda al futuro con serenità e con pragmatismo: pragmatismo: abbiamo parlato anche dei pirati del Mar Rosso e l'obiettivo è quello di creare strumenti di coordinamento e cooperazione a livello di G7 che siano in grado di aumentare il livello di preparazione in risposta alle crisi e agli *shock*

(penso all'Ucraina): ricostruire con guerre in corso è infatti assolutamente complicato, quindi mi auguro che tutti coloro che hanno responsabilità di governo tornino a costruire ipotesi e percorsi di pace e non preparino

agricole, mentre mettere fuori norma e fuori mercato dal 2035 le auto o le moto a diesel e benzina è una follia priva di qualsiasi senso); il ruolo centrale dell'industria, che va coinvolta nella transizione; l'importanza di seguire un approccio globale, anche in settori come anche quello marittimo e dell'aviazione, perché la decarbonizzazione non può essere pagata esclusivamente dalle imprese e dai cittadini. Come ha detto il ministro Giorgetti, chi paga? Non si imporre una nuova tassa sulla casa e il cambio della macchina; poi in alcune città - permettetemelo, da milanese - vietare l'ingresso ad alcune migliaia di motociclisti è assolutamente un controsenso: ringrazio infatti chi usa le due ruote, perché contribuisce a snellire il traffico e inquinare di meno. In sostanza, questo G7, partendo da Milano e dall'Italia, con politiche di buon senso e non ideologiche, pensa a un futuro e a un ambiente più puliti e alla decarbonizzazione. Il mio obiettivo, però, da vice presidente del Consiglio e avere un'Italia sicuramente più *green*, ma non totalmente disoccupata, perché sarebbe il fallimento. perché, oltre a evidenziare le risultanze del G7, sottolinea una posizione ben chiara da parte del Governo: quella di perseguire

soprattutto per quanto riguarda gli investimenti nel settore dei biocarburanti, che potrebbero portare proprio alla neutralità tecnologica, capace di tutelare l'ambiente, ma contestualmente senza ripercussioni economiche e anche occupazionali. Crediamo in uno sviluppo sostenibile, in grado di trovare un nuovo equilibrio tra natura e uomo. La sostenibilità non può ridursi a una mera dichiarazione di intenti. Per questo c'è la necessità di affiancare alla sostenibilità ambientale anche quella economica, come lei ha ricordato quest'oggi in Aula. La sfida che ci attende nel futuro è proprio quella di far coesistere la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica con l'esigenza della società di innovarsi e del tessuto economico di continuare

anni fa la legge n. 508 del 1999 ha previsto la trasformazione delle accademie e dei conservatori in istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Da allora doveva partire un progetto di norme e di regolamenti per rendere organico il sistema. Alcune cose sono state fatte in questi venticinque anni, alcuni regolamenti sono stati adottati; il sistema è ancora molto disomogeneo, non è assolutamente

investimento sul futuro perché queste sono istituzioni che per il nostro Paese, per la nostra cultura, rappresentano un investimento per il futuro. Alla luce di tutto questo, le chiedo, Ministro, se

Senatore Damiani, per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - detta AFAM - siamo riusciti a portare a compimento misure che - come lei ha giustamente ricordato - erano attese da molti anni, certamente almeno venticinque. E per questo ringrazio lei e con lei tutto il Gruppo Forza Italia, il capogruppo, presidente Gasparri, che vedo presente in Aula, perché mi offre l'occasione di riferire al Parlamento intero sul lavoro che stiamo facendo per un settore che - come ha detto giustamente lei - rappresenta un grande investimento sul futuro del nostro Paese; un elemento di grande innovazione non solo di migliore tradizione artistica e culturale, ma anche di grande innovazione e di grande prospettiva futura. Certamente è una finestra sul mondo delle bellezze presenti e future del nostro Paese. Dalla mia presa di servizio, l'Alta formazione artistica è stata una priorità non solo a parole e quanto fatto direi ne è una dimostrazione palmare. Martedì scorso - per ricordare le ultime determinazioni acquisite in questo ambito - abbiamo approvato in Consiglio dei ministri il regolamento sul reclutamento del personale docente, quello a cui faceva riferimento, per dare un inquadramento, uno *status* con carattere di definitività al personale docente e tecnico-amministrativo degli istituti AFAM. Unitamente a quello sul personale docente e tecnico-amministrativo, abbiamo anche approvato il regolamento sugli ordinamenti didattici. il reclutamento, mettiamo le basi per la costruzione di un sistema omogeneo, in grado di assicurare una più alta qualificazione professionale, introducendo l'abilitazione artistica nazionale, similmente a quanto già avviene come Alta formazione per il sistema universitario; un ulteriore passo verso quella equiparazione dei due sistemi, non formale ma sostanziale così significativamente e direi senza interruzioni invocata dalla categoria. Con la riforma degli ordinamenti didattici rendiamo l'insegnamento più flessibile e interdisciplinare, ma anche più specialistico, ampio, innovativo. Finalmente diamo vita alla figura del ricercatore AFAM, una novità estremamente importante nel segno dell'autonomia di istituzioni che da sempre fanno ricerca, ma che ora viene finalmente e giustamente riconosciuta. Sono misure nelle quali crediamo moltissimo e che abbiamo fortemente voluto, ma che non esauriscono il nostro lavoro. Stiamo già ultimando altri due regolamenti, uno sulla programmazione e valutazione della qualità della ricerca e un altro sulla *governance*. Sono azioni, non annunci, che dimostrano quanto per noi l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sia strategica, un elemento portante del nostro sistema di infrastrutture creative, perché queste sono infrastrutture immateriali che il mondo ci richiede e verso cui il mondo viene, ma anche un veicolo culturale e identitario, capace di intercettare il desiderio, diffuso ovunque, di avvicinarsi al nostro Paese e alla nostra cultura.

anche per quanto riguarda la mia Regione, la Puglia, molto interessata da queste istituzioni. Rispetto alle criticità che ho elencato nel primo intervento e nella domanda soddisfatto perché mi rendo conto che già sul reclutamento del personale sono stati adottati dei regolamenti e quindi abbiamo già superato questa criticità, come anche con tutta la riforma organica cambia la didattica, che diventa più flessibile e interdisciplinare e quindi si garantisce un'offerta migliore anche agli studenti, un'altra criticità

Ricordo anche, perché abbiamo esaminato qui la manovra finanziaria, di cui sono stato anche relatore, i 200 milioni da investire sul patrimonio immobiliare di queste istituzioni. Ringrazio il Ministro per la risposta e la invito a continuare ad investire su queste istituzioni, perché sono il fiore all'occhiello del nostro Paese.

Ho letto che già solo per aver espresso qualche preoccupazione e qualche dubbio si parla di guerra alle università telematiche. Noi pensiamo che invece sia davvero un fenomeno a cui guardare con grande attenzione.

Cambia anche l'età delle persone che si iscrivono alle università telematiche: sempre di più sono giovanissimi, che hanno meno di ventitré anni, quindi si scrivono direttamente dalla maturità. Sempre meno le università telematiche rispondono ai bisogni degli studenti universitari o al recupero di anni per persone che avevano magari lasciato Tutto questo avviene in università che hanno un personale di ruolo ridotto, un rapporto docenti-studenti molto inferiore a quello esistente nelle università tradizionali, talvolta una totale assenza di strutture di ricerca, cose che pregiudicano la possibilità di seguire anche l'attività formativa in modo corretto e c'è un tema serissimo di accreditamento, di *standard* qualitativi, in materia di autovalutazione, di valutazione, di accreditamento iniziale e periodico, delle sedi sedi e dei corsi di studio e questo ce lo dicono i dati. Quello che le chiediamo è come viene fatto il monitoraggio dell'adeguamento di queste università agli *standard* richiesti dal decreto del 2023. Teniamo presente che c'erano anche forze politiche che hanno provato a rimandare ulteriormente questo adeguamento e ci risulta che la gran parte degli esami avvengono *online*, mentre non sarebbe possibile per le università telematiche fare questo, secondo la legge del 2003 che le disciplina. Ministro su quali norme state ragionando al fine di assicurare una più rigorosa ed efficacia regolamentazione di questo sistema.

è - lo ha ricordato e ha ragione - molto importante. È un tema su cui ci stiamo misurando molto. Faccio una premessa alle risposte che poi le darò: è un tema talmente importante che avverto molto la ristrettezza dei tempi di un *question time*, però mi riservo di parlarne più approfonditamente magari in altra sede, sempre però da condividere in ambito parlamentare. Le università telematiche sono una realtà: sono e offrono percorsi formativi sia interamente a distanza, sia parzialmente a distanza. Sono atenei che costituiscono un tassello ormai definito. Lei ha ricordato l'aumento esponenziale di tali università. Questo ci dice due cose: primo che esistono; secondo che intercettano un bisogno che anche le università tradizionali

anche - sottolineo - a distanza. Il Covid ci ha aiutato a fare un passo in avanti sia nelle comunicazioni, sia nella didattica, nella qualità dell'offerta formativa. Le università in presenza hanno organizzato iniziative di didattica a distanza; alcune stanno proseguendo, altre no. Questo significa che prima di tutto le università telematiche non sono un pezzo di mondo universitario che si muove in un *far west* di assenza di regole e controlli. I percorsi di studio delle università telematiche sono decisamente controllati e accreditati dal Ministero che mi onoro di rappresentare e soprattutto soggetti, come le altre università, come le università in presenza, alla valutazione dell'ANVUR, che è l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ha citato alcune disposizioni, alcune di normazione secondaria che hanno ridisciplinato i meccanismi di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale periodico delle università telematiche. Questo è il senso: le università in presenza e le università telematiche devono avere la stessa modalità di regolamentazione, tenendo conto delle specifiche di contesto. La didattica in presenza non è come la didattica a distanza (purtroppo sto già

un tavolo di lavoro che ricomprende le università telematiche la Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e l'ANVUR, in cui stiamo dando regole comuni a tutte le università in modo da fare l'unica cosa che il Ministero deve assolutamente fare: garantire la qualità dell'offerta formativa a tutti, per tutti, con ogni modalità di erogazione dell'offerta didattica. Il Ministero dell'università non è l'Antitrust, non deve regolare i rapporti tra università telematiche o tra università telematiche e università in presenza; deve fare una cosa fondamentale, che è quella che ci impegniamo a fare con tutte le nostre forze: garantire, a vantaggio delle studentesse e degli studenti, la qualità dell'offerta formativa. Gli esiti di questo tavolo - a questo saranno mirati - ricomprenderanno sia le università in presenza, sia le università a distanza, calcolando che il modello verso cui stiamo andando è un modello *blended* (misto), dove, per esigenze che evidentemente si manifestano per i numeri che lei ha giustamente evidenziato, anche le università in presenza devono dare risposta a questo ambito di richiesta. PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice D'Elia, per due minuti. Signor Presidente, ringrazio la Ministra per la risposta. Sicuramente ci saranno altre occasioni e torneremo sull'argomento, ma non posso dirmi soddisfatta, perché è vero che si intercettano bisogni, ma il tema è anche questo. che, in assenza di un *welfare* studentesco forte e di questioni di diritto allo studio non risolte in questo Paese, su cui stiamo discutendo, che riguardano anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli alloggi e le residenze, la scorciatoia

Ancora, nelle dovute differenze, noi abbiamo bisogno che le regole siano veramente applicate. Sono emerse troppe criticità riguardanti le università telematiche. Citavo il caso degli esami, che andrebbero fatti comunque sempre in presenza. Queste università sono diventate società di capitali, sono state sono state acquistate da fondi di investimenti stranieri. C'è un tema riguardante il profitto, che può confliggere con la qualità della didattica, e su questo noi dobbiamo assolutamente vigilare.

*(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi, per l'ennesima volta, sono ancora in quest'Aula a parlare di autonomia differenziata, e dal ministro Calderoli a tutti i quesiti posti non è seguita una parola. Mi chiedo se non sia una strategia. No: non sa cosa dire ed egli stesso è consapevole dello scippo che le ricche Regioni del Nord stanno attuando a danno delle Regioni del Sud. l'autonomia differenziata è lo strumento inventato dalle Regioni più ricche del Paese per tentare di tenersi quasi interamente l'importo delle tasse che spettano all'Italia intera. La cosa grave è che il Governo ha depennato dai fondi del PNRR sedici miliardi di risorse destinate al Sud e nell'ultima legge di bilancio ha sottratto ai Comuni fragili diversi miliardi dal Fondo di solidarietà comunale. Inoltre, ha sforbiciato quattro miliardi dal Fondo perequativo infrastrutturale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi giorni ho avuto un lungo confronto con il professor Massimo Villone,

al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie. Inoltre, come disciplinato dall'articolo 11, comma 1, gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge. Ciò significa che potrebbero essere riprese le carte già preparate tra il 2018 e il 2019 con le tre Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Alla luce di queste due disposizioni e a seguito del colloquio col professor Villone, ho redatto un'interrogazione in cui chiedo al Governo: di conoscere i limiti richiamati dall'articolo 2, comma 2, che si intendono porre al negoziato con le Regioni per la tutela dell'unità giuridica ed economica e delle politiche prioritarie per il Paese; di conoscere l'orientamento verso possibili iniziative di coordinamento tra Regioni in chiave di macroregione; di conoscere quali e quante, delle 184 e più funzioni richiamate nelle intese già presentate al Governo, siano in concreto immediatamente trasferibili. signor Presidente, onorevoli colleghi, come saggiamente rimarcato dal professor Villone, al fine di tutelare l'unità del Paese, a seguito dell'approvazione di ulteriori forme di autonomia le Regioni meridionali hanno il dovere civico e politico di depositare presso la Corte costituzionale un ricorso avverso la legge Calderoli. Io sono impegnata, con tutti i colleghi del MoVimento 5 Stelle, a sollecitare i Presidenti delle Regioni meridionali ad agire presso la Corte il giorno dopo l'approvazione di questa legge. legge. Solo così sarà possibile sperare ancora in un Paese unito e coeso, come dettato dalla normativa europea, all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dalla nostra Carta costituzionale.